Comunico che in data 1° ottobre 2024 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia:* «Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni, nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria»

è completamente paralizzato per un guasto. È l'ennesimo episodio che segue un'estate di enormi disagi per tutti gli utenti del sistema ferroviario italiano.

pertanto al ministro Salvini di venire in Senato e, una volta per tutte, spiegare al Parlamento e agli italiani che cosa ha intenzione di fare per affrontare una situazione intollerabile e indegna di un Paese civile. Andate nelle stazioni e verificate di persona che cosa sta succedendo e quanti colleghi, peraltro, sono bloccati e non riescono a venire a causa di quanto successo oggi al nodo di Roma, ma che segue decine e decine di interruzioni che hanno costellato l'estate di milioni di italiani.

Dal Ministro ancora nessuna risposta. La cosa è incredibile e non è possibile continuare di questo passo. Per questo appoggiamo la richiesta del collega.

È indispensabile che il Ministro renda conto al Parlamento di quello che sta succedendo, perché stiamo arrivando a livelli insostenibili. Oggi qualcuno scriveva sui *social* non c'è niente di peggio di un Frecciarossa che parte con un'ora e mezza di ritardo e di un Frecciarossa delle 6,30 del mattino che parte con un'ora e mezza di ritardo. Aggiungo che, quando si arriva alla stazione Termini, l'eventuale risparmio di tempo dovuto all'Alta velocità si passa aspettando un taxi, naturalmente, senza una pensilina, sotto il sole e sotto la pioggia, per un'ora. Quindi, non funziona più niente. Ripeto: almeno quando c'era lui i treni arrivavano in orario; adesso no.

vi prometto che farò un elenco delle giornate e di quante ore perdiamo in treno, perché davvero i treni non funzionano. Addirittura treni che partono da Milano

poche balle da questo punto di vista e vediamo di affrontare il tema.

legittimo, di fronte a un guasto della rete ferroviaria con difficoltà e problematiche che riguardano alcune stazioni importanti, *in primis* quella di Roma, chiedere un'informativa al Ministro per capire la situazione delle reti, è giusto che il Parlamento sappia quali sono gli investimenti che il Ministero vuole fare per potenziare la rete e migliorare il servizio ai cittadini. Ci Ci mancherebbe altro e c'è da parte nostra un certo disagio nel vedere che i cittadini sono ovviamente in difficoltà per quello che è accaduto.

per strumentalizzare la vicenda e attaccare il ministro Salvini, come se fosse responsabile della manutenzione delle reti ferroviarie che c'è stata negli anni con dei Ministri che non sono stati del centrodestra è davvero uno scandalo *(Proteste)*! È una vergogna che si utilizzino questi episodi per attaccare una maggioranza e un Ministro! Soprattutto, questo dà la dimensione del livello basso in cui l'opposizione si è ridotta negli ultimi tempi: senza idee, senza progetti e solo strumentalizzando qualsiasi guasto possa accadere. Vergognatevi! Vergognatevi! Vergognatevi!

CAPARVI ed altri. -*** ***Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*** Il relatore, senatore Speranzon, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi Presidente, onorevoli colleghi, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 1038, recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. La 7a Commissione permanente ne ha concluso l'esame in sede redigente lo scorso 8 maggio, senza apportare modifiche al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Il disegno di legge, a prima firma dell'onorevole Caparvi ed altri, si compone di 12 articoli suddivisi in tre capi. Il capo I (articoli da 1 a 9) reca disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica. L'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale della Nazione ed elementi qualificanti per la formazione e la crescita socioculturale della comunità nazionale. L'articolo 2 reca le definizioni di ente di rievocazione storica e di manifestazioni di rievocazione storica. L'articolo 3 dispone circa le attività promosse dallo Stato nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate a riconoscimento, sostegno, valorizzazione e salvaguardia delle specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socioculturali regionali e locali ad esse collegate. L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, di un elenco nazionale avente funzione ricognitiva degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica. A tal fine si autorizza la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dal 2024. La definizione dei requisiti per l'iscrizione all'elenco e delle relative modalità di gestione è demandata a un decreto ministeriale. L'articolo 5 prevede l'istituzione, da parte del Ministero della cultura, di un comitato tecnico-scientifico, al quale è affidato il compito di riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica e di fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche. Al comitato sono attribuiti altresì compiti di ricerca, studio, formazione e aggiornamento in materia. L'articolo 6 stabilisce che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, approvi ogni anno l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo dandone ampia diffusione. L'articolo 7 concerne le iniziative didattiche nelle scuole finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti. L'articolo 8, proponendo novella alla legge n. 110 del 1965, consente ai partecipanti alle manifestazioni in esame l'esibizione, il porto e l'uso di armi da fuoco fabbricate anteriormente al 1950 (o loro repliche) con munizioni a salve, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Alle medesime condizioni è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti. L'articolo 9 reca disposizioni relative all'accensione di fuochi nelle manifestazioni in oggetto e nelle ricorrenze della tradizione popolare. Il capo II in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale si compone degli articoli 10 e 11. prevede, tra l'altro, che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale. L'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale in conformità alle disposizioni della Convenzione UNESCO in materia. Sono quindi dettagliati i principi e i criteri direttivi della delega. L'articolo 12, unico articolo del capo reca la clausola di salvaguardia, che rende applicabili le disposizioni in esame nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti».

si intendono illustrati.

Prego, senatrice. Adesso c'è abbastanza silenzio. proposta, mi preme sottolineare un aspetto politico. Questa mattina - e anche nei giorni scorsi stiamo vivendo una situazione difficilissima, complicata, prima di tutto per quello che sta accadendo in Medio Oriente, con le Commissioni esteri e difesa riunite fino a poco fa,

Allora io vi chiedo come si fa - e potrei continuare con altri temi che interessano la vita quotidiana dei cittadini - a non dare priorità a questi temi e a non avere il Governo in Aula,

non si può tacere rispetto a una situazione difficilissima, con notizie che arrivano di ora in ora, soprattutto sul conflitto in Medio Oriente, che ci preoccupano davvero

certamente favorevoli dal punto di vista del valore storico, ma anche - aggiungo - turistico che questo provvedimento avrà poi a cascata sui territori. Parto dall'aspetto storico, perché conosciamo tutti la storia che viene studiata nelle nostre scuole. È però altrettanto importante sottolineare, ricordare e avere memoria storica degli aspetti - qui sì - storici a livello locale. Per questo dobbiamo ringraziare gli enti locali per quello che ogni anno riescono a fare nei loro territori, ormai senza risorse economiche, grazie al lavoro appassionato dei volontari, a cui va un ringraziamento anche da questo Senato. Non possiamo però non ricordare che quelle manifestazioni ormai vivono grazie al contributo del volontariato e delle tante persone che ancora credono e vogliono mantenere un'identità, vogliono parlare e ricordare le loro radici storiche. Ricordo a quest'Assemblea che le rievocazioni storiche riguardano oggi più di 1.300 eventi su 8.000 Comuni

importante perché la passione, l'identità che viene ricordata attraverso dette manifestazioni ci ricorda anche dal punto di vista turistico, il patrimonio immobiliare è stato riconosciuto con la Convenzione dell'Unesco nel 2003. Si tratta di un riconoscimento importante che non dobbiamo dimenticare e che deve essere visto non come un traguardo, ma come un punto di partenza proprio per il valore turistico, culturale e storico che tali manifestazioni hanno. quindi di una congiunzione importante tra storia e turismo.

Chiediamo però al Governo che ci siano, oltre all'impegno degli enti locali, anche un impegno e un coinvolgimento delle scuole e l'utilizzo tecnologico e informatico per far conoscere la storia dei nostri eventi territoriali storici. ricordare però, anche da questo punto di vista, che queste manifestazioni storiche devono avere un riconoscimento che vada oltre l'Italia, un riconoscimento, appunto, a livello europeo, perché è la storia, il patrimonio culturale dell'identità stessa della nostra Nazione. Vado a chiudere, dicendo che credo che da questo punto di vista sicuramente ci sarà

meno slogan e più impattanti anche dal punto di vista valoriale, identitario ed economico.

Signora Presidente, la tutela delle manifestazioni rievocative ha a che vedere con la conservazione della memoria del passato, ma ha anche ripercussioni sul settore turistico e culturale di un determinato territorio e, non di rado, è l'occasione per raccogliere fondi di solidarietà e di beneficenza. Sono tantissime le realtà associative che nascono intorno alle manifestazioni, riuscendo ad accomunare persone che altrimenti, spesso, avrebbero poco in comune. Il folklore e le tradizioni trascendono infatti le appartenenze politiche, ideologiche o religiose e vedono coinvolte fianco a fianco persone di qualsiasi ceto sociale, e questo ci piace molto. Questa ricchezza che contraddistingue tante realtà nel nostro Paese va tutelata. Le rievocazioni storiche permettono anche a chi arriva da un altro luogo, da un altro Paese, da un'altra cultura di inserirsi dentro le comunità del luogo e conoscere la cultura che li ospita. Cos'è oggi la comunità locale, se non l'incontro tra culture e tradizioni diverse? È quella commistione che si arricchisce nel vivere e, nel caso dei bambini, anche nel crescere insieme. Ci sarebbe piaciuto, Presidente, che questa proposta di legge avesse qualche attenzione in più all'aspetto dell'intercultura e della creazione di comunità nel territorio. Ma confidiamo che una tale mancanza possa essere colmata nelle articolazioni della proposta di legge che vede il coinvolgimento delle scuole - queste per loro stessa natura, attrezzate per la partecipazione di tutte le bambine e di tutti i bambini, di tutte le ragazze e di tutti i ragazzi. Signora Presidente, nonostante questi aspetti positivi, devo dire che, per tutelare le manifestazioni e le rievocazioni storiche, si sia dovuti ricorrere a una proposta di legge, quando sarebbe bastato probabilmente un provvedimento del Ministro, e non necessariamente l'impegno di questo Parlamento per ore ed ore. Lo diciamo perché capita sempre più spesso di trovarsi in questa situazione: al Governo fanno decreti-legge sulle cose importanti del Paese, da quelle economiche a quelle sociali. Quindi, di fatto, determinano tutta la discussione sulle cose fondamentali all'interno dei palazzi del Governo, per poi venire qui a mettere la fiducia. Nel frattempo si tiene impegnato il Parlamento a discutere di temi e questioni che pure ci stanno a cuore - lo ribadisco - ma sono laterali rispetto alla centralità di quelli che toccano la vita di tutte le cittadine e di tutti i cittadini. Sarebbe più facile, invece, fare il contrario: dare ai Ministeri il compito di seguire e tutelare in questo caso la realtà delle rievocazioni e delle manifestazioni storiche, anche finanziandole, laddove lo si ritiene opportuno - noi in molti casi lo riteniamo opportuno e permettere invece al Parlamento di discutere dei temi un po' più ampi e un po' più larghi, che riguardano la vita materiale di tanti e tante che oggi si trovano in serie difficoltà. Per cui, signora Presidente, noi voteremo a favore di questa proposta di legge. E lo faremo perché ci stanno a cuore queste iniziative territoriali, perché le troviamo belle e molto spesso sono elementi che arricchiscono la vita dei cittadini, troppo spesso minacciata dalla solitudine, che è una delle grandi caratteristiche del tempo in cui viviamo.

colleghe e colleghi, quando pensiamo alla cultura è facile che ci vengano in mente monumenti, opere d'arte e architetture imponenti, ma la verità è che il cuore pulsante di una civiltà risiede in quello che non si vede, nella sua anima, nelle tradizioni, nei gesti, nei racconti che attraversano le generazioni. Sono queste memorie intangibili che nel tempo modellano la nostra identità collettiva. Durante i miei studi di architettura ho imparato una lezione fondamentale: prima di progettare qualsiasi spazio, è necessario ascoltare il *genius loci*, lo spirito del luogo. Questo concetto antico ci insegna che ogni territorio ha una sua anima, qualcosa che va oltre ciò che è visibile: è l'atmosfera che si percepisce camminando tra le strade di un borgo, partecipando a una festa tradizionale o ascoltando una vecchia storia raccontata dagli anziani. Questo spirito si manifesta non solo attraverso gli edifici, ma anche e soprattutto attraverso le tradizioni, i riti, le memorie che da secoli plasmano quel contesto. Il disegno di legge in discussione tocca proprio questo tema: le manifestazioni storiche e la salvaguardia del patrimonio immateriale. Rievocare la storia di un luogo significa non solo guardare al passato, ma anche risvegliare quel *genius loci* che lo rende unico, dando vita a ciò che è invisibile, ma profondamente presente. Pensiamo per un attimo alla civiltà romana: certo, il Colosseo e il Pantheon sono icone che ammiriamo ancora oggi, ma ciò che ha reso grande Roma non è solo la pietra, sono la *lex romana,* le tradizioni civiche e religiose, l'organizzazione dello Stato e quella sociale che hanno plasmato la vita di ogni cittadino, di ogni *cives*. Questi sono gli aspetti immateriali che hanno resistito ai secoli più di qualsiasi monumento. Sono quei valori invisibili che hanno dato forza e coesione all'impero. ciò che ci rimane impresso non sono solo i monumenti, ma anche una serie di sensazioni profonde: sono i suoni, i profumi e i colori; sono soprattutto le esperienze quelle che ci toccano nell'intimo. Nel corso di più di dieci viaggi in Cina ho potuto ammirare grandi monumenti, come la Città proibita e la Grande muraglia, ma a restarmi impressi sono stati gli elementi di vita quotidiana, tradizioni e ritualità che permeano quella cultura cinese. I monaci Shaolin, per esempio, sono figure emblematiche della cultura cinese, custodi di una tradizione millenaria che combina arti marziali e meditazione. Osservare la loro disciplina la ricerca della perfezione nei movimenti è stato come toccare con mano una delle espressioni più profonde della cultura immateriale cinese: l'armonia tra corpo e spirito, tra individuo e natura. Ci sono scene collettive anche per strada in Cina: sono apparentemente semplici esercizi fisici, che invece rappresentano una lunga tradizione di benessere condiviso. Nei parchi e nelle piazze, il *tai chi* e le altre pratiche simili non riguardano solo la salute del corpo, ma anche l'equilibrio mentale e spirituale; sono riti quotidiani che trasformano un luogo in uno spazio di benessere collettivo. È un esempio perfetto di come la cultura immateriale e il benessere olistico possano essere vissuti quotidianamente nella comunità. Questi aspetti, fatti di tradizione e di gesti quotidiani, sono ciò che davvero si imprime nella memoria, non sono solo monumenti di pietra o grandi opere architettoniche, ma esperienze che ci connettono al *genius loci* di un luogo, alla sua essenza più profonda. Mi sono soffermato su questa mia esperienza personale per testimoniare come il patrimonio immateriale sia ciò che fa sì che un luogo non sia semplicemente uno spazio geografico, ma anche un'esperienza culturale viva: è ciò che trasforma un monumento in qualcosa di significativo, che dà valore e anima alle pietre. Senza memoria, senza storia, senza tradizioni, i monumenti diventano gusci vuoti. Sono le attività immateriali che danno significato ai nostri luoghi. Pensiamo per un attimo al fuoco olimpico, un simbolo che risale ai tempi greci, che è fatto non di pietra o metallo, ma di luce e di spirito, e, ogni volta che viene acceso, il mondo intero si raccoglie attorno ai valori di fratellanza, competizione, e pace. Una fiamma arde nel cuore della comunità, alimentando la memoria e il senso di appartenenza. Anche la «Divina Commedia» non è solo un capolavoro letterario, ma è anche una riflessione profonda sull'eredità culturale del popolo. Dante, nel suo viaggio attraverso i tre regni dell'aldilà, porta con sé la memoria della della cultura classica e cristiana, mostrando come il passato sia indispensabile per comprendere il presente e il futuro. Le rievocazioni storiche, le tradizioni orali, le botteghe artigiane non sono semplici spettacoli: sono memoria vivente. Pensiamo alla commedia dell'arte o alle grandi manifestazioni come il Palio di Siena o la Regata storica di Venezia: ogni anno queste tradizioni attirano migliaia di visitatori, dimostrando che il nostro patrimonio immateriale è anche un motore per l'economia e per il turismo culturale. Il valore di questo disegno di legge è nel riconoscere che queste tradizioni sono non solo eredità del passato, ma risorse vive per il nostro presente e per il futuro; non possiamo permettere che scompaiono o che diventino semplici oggetti da museo, ne devono rimanere nelle mani e nei cuori delle persone. Il coinvolgimento della comunità è essenziale: le nostre tradizioni devono essere vissute e mantenute vive e il nostro compito è sostenerle, non solo conservandole, dando loro spazio per crescere. Così come un grande edificio ha bisogno di essere vissuto, anche la cultura immateriale deve fiorire. Questa legge non solo riconosce il valore del nostro patrimonio immateriale, ma promuove gli enti locali, che sono i veri custodi di queste tradizioni. Inoltre, la promozione della cultura ha un impatto economico significativo: ogni euro speso in cultura ha un moltiplicatore importante sul PIL e, poiché molte di queste manifestazioni sono alimentate dal volontariato, l'impatto economico è ancora maggiore. signor Presidente, Forza Italia esprime il proprio voto favorevole. Siamo qui non solo per approvare una legge, ma anche per riconoscere e valorizzare ciò che spesso sfugge agli occhi, ma non al cuore, è quello che dà profondità e anima ai nostri luoghi, alle nostre vite, alle nostre comunità. Custodirlo è non solo un atto di protezione, ma anche un atto di fiducia nel futuro. Se le pietre possono crollare, se i monumenti possono essere distrutti, la memoria e le tradizioni restano vive finché ci saranno persone pronte a viverle e a tramandarle. Quello che facciamo qui è non solo proteggere il passato, ma dare continuità a una storia che ci lega e ci proietta verso il domani. Non è la semplice tutela di un'eredità, l'impegno a farla crescere, ad alimentarla, a renderla parte viva della nostra quotidianità. *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella più famosa affermazione del suo testo «Prediche inutili», Luigi Einaudi, grande economista e seconda Presidente della Repubblica italiana, poneva una domanda che ancora oggi è fondamentale per ogni buon legislatore: come si può deliberare senza conoscere? La sua risposta era netta: è impossibile. Dunque, è innegabile che la nostra memoria storica e le manifestazioni che la celebrano siano essenziali per la costruzione e la crescita dell'identità di una comunità. Le rievocazioni storiche, infatti, non solo ci permettono di riscoprire il nostro passato, ma fungono anche da catalizzatore per la coesione sociale e strumenti per l'educazione delle nuove generazioni. Esse sono parte integrante del nostro patrimonio immateriale, così come lo sono, ad esempio, le lingue dialettali. Pertanto, il MoVimento 5 Stelle non remerebbe mai contro un testo che intende valorizzare uno degli *asset* della nostra terra. Tuttavia, l'idea di un patrimonio culturale immateriale non può e non deve diventare un mero strumento di *marketing*, tanto caro a questo Governo "Dio, Patria, Famiglia", per eventi che non hanno realmente un legame con la nostra storia. Certo, leggendo il provvedimento, apprendo all'articolo 5 che avete pensato di istituire un comitato scientifico incaricato di riconoscere la qualifica di ente e di manifestazione di rievocazione storica. Mi chiedo l'ennesimo consesso di potere alimentato da un Esecutivo che, da inizio legislatura, si sta dilettando nel consegnare poltrone e ruoli, così da accrescere il cerchio di potere del Governo, quando certamente si sarebbe potuta ampliare la già esistente procedura ministeriale per i beni mobili e immobili prevista dal nostro codice per i beni culturali all'articolo 12 e seguenti. Apprendiamo, poi, che questa misura prevede per questa iniziativa un sostegno statale generico non quantificato e, quindi, una vera scatola vuota. È innegabile che stiamo pur sempre parlando dell'Esecutivo della propaganda e, dunque, dell'ennesimo provvedimento senza fondi. Mi viene da sorridere leggendo, ad esempio, l'elenco delle finalità cariche di buone intenzioni previste dall'articolo 3. Riporto testualmente tale articolo: «Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali a queste collegate». Così recita in pompa magna il comma 1, rafforzando il messaggio alla lettera *d)* del medesimo articolo, dove si sostiene di voler sostenere finanziariamente gli enti di rievocazione storica e la realizzazione delle relative manifestazioni nonché gli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi, attraverso idonee misure. Onorevoli colleghi, è facile immaginarsi lo stato di euforia di chi lavora in questo settore, di quanti, leggendo queste righe, saranno portati a pensare che finalmente il Governo è in procinto di sostenere economicamente questo settore culturale. La verità però è tutt'altra ed è veramente amara. Approfondendo il provvedimento e decodificando quei tecnicismi che possono risultare ostici ai non addetti ai lavori, viene infatti fuori un'altra verità, e cioè che le risorse saranno a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, da destinare alle rievocazioni stesse. Ciò significa che l'Esecutivo vuole far credere che verranno destinate ulteriori risorse, salvo poi menzionare un capitolo del bilancio statale dedicato a questo tipo di attività, che già esiste e già viene utilizzato da tempo. Se però il Governo realmente avesse voluto supportare le rievocazioni storiche, avrebbe dovuto stanziare una dotazione aggiuntiva e non citare un fondo vecchio e sottodotato. verità allora è un'altra, e cioè che le uniche risorse stanziate, previste dall'articolo 4 per il mantenimento dell'elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica, ammontano a 10.000 euro. Sì, avete capito bene, onorevoli colleghi: sono stati stanziati appena 10.000 euro, un importo che probabilmente non riesce nemmeno a coprire le spese per un pony da far sfilare al Palio di Siena. Diversi dubbi si annidano anche nell'articolo 8, che disciplina il porto e l'uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, e nell'articolo 9, che norma l'accensione di fuochi nelle manifestazioni di rievocazione storica e nelle ricorrenze della tradizione popolare. Sebbene comprenda l'importanza delle tradizioni folcloristiche, che fanno piacere anche a me, per noi legislatori è fondamentale considerare la sicurezza dei cittadini e il messaggio che stiamo inviando. I due articoli citati presentano purtroppo numerosi profili di criticità, che meritano una riflessione approfondita. La presenza di archi, balestre, spade e altri strumenti da combattimento rischia di inviare un messaggio confuso. Infatti, da un lato, celebriamo la storia e le tradizioni e, dall'altro, sembrerebbe legittimare e mitizzare l'uso di armi come parte della nostra cultura nella mente dei più piccoli.

Onorevoli colleghi, non è mia intenzione o meglio non voglio mettere in dubbio la preparazione di chi, nel corso delle nostre manifestazioni storiche, maneggia le armi a salve, ma faccio una considerazione. Mentre difficilmente archi e balestre possono accidentalmente colpire qualcuno, non si può dire altrettanto per le armi da fuoco. Inoltre, le Forze dell'ordine, già oberate da compiti di vigilanza e controllo su fenomeni ben più gravi, sarebbero ulteriormente gravate dal compito di monitorare eventi che per loro natura dovrebbero essere occasione di festa e convivialità. Come se non bastasse, l'accensione di fuochi durante queste manifestazioni rappresenta un ulteriore fattore di rischio. Infatti, non solo la gestione del fuoco richiede competenze specifiche e precauzioni rigorose, ma il potenziale per incidenti è alto, soprattutto in contesti affollati. Le tradizioni possono e devono essere onorate in modi che non coinvolgono elementi di violenza o di potenziale pericolo. Vorrei evidenziare inoltre una problematica normativa che potrebbe derivare dall'articolo 11. Certo, sono perfettamente cosciente del fatto che la nostra normativa vigente presenta una carenza dal punto di vista della gestione del patrimonio immateriale, nonostante la ratifica della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, della successiva Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, ai sensi della legge 1° ottobre 2021, n. 133. Entrambe risultano insufficientemente assorbite dall'articolo 7-*bis* del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Effettivamente il nostro testo unico risulta carente sui beni immateriali, ad eccezione del paesaggio.

del nostro patrimonio culturale immateriale, fatto non solo di sfilate storiche, ma di lingue, testi, canzoni, fiabe, filastrocche *et similia*, lo trovo a dir poco sconcertante. Leggo infatti testualmente, al comma 3 dell'articolo 11, che i decreti legislativi andranno ad abrogare espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali. Onorevoli colleghi, parliamo quindi di un cambiamento che potrebbe essere estremamente impattante sulla normativa vigente e che avrebbe necessitato di un ampio dibattito preliminare in ambito parlamentare. Ma questo non è avvenuto. Pertanto, seppur per certi versi favorevoli, almeno parzialmente, all'iniziativa, le nostre perplessità non ci consentono di esprimerci in maniera favorevole e quindi ci asteniamo.

ha visto fiorire modi di pensare e di fare, usi e costumi, tradizioni tanto varie e diverse. In Italia non è mai esistito, come in altre Nazioni, un centro politico e culturale unificatore, un luogo deputato più di altri a elaborare modelli culturali da irradiare poi in periferia; non sono esistite culture e tradizioni omogenee dominanti. L'Italia, infatti, è la terra dei comuni medievali e delle signorie rinascimentali, dei mille campanili, degli antichi borghi, della sana e vitale competizione fra località vicine geograficamente, eppure ognuna tesa a superare l'altra in bellezza e creatività. La diversità La diversità ha costituito la cifra della nostra cultura, la fonte che l'ha resa unica e inconfondibile, ricca quanto nessun'altra al mondo. La diversità è anche la caratteristica principale della nostra identità, che è plurale per definizione. Tocca a noi preservare, conservare, promuovere e valorizzare questa identità, ovvero questa ricchezza e varietà culturale sedimentatesi non solo nei beni materiali, quali le opere d'arte e i monumenti di cui sono pieni tutti i luoghi della nostra penisola, ma anche nei beni immateriali e rappresentati dalle tradizioni che si sono trasmesse di generazione in generazione, arrivando fino a noi. È un'operazione tanto più urgente e necessaria in un mondo, come quello di oggi, in cui i processi di globalizzazione tendono a favorire l'omogeneità e l'omologazione e a far scomparire le identità locali in una cultura unica e standardizzata. Lo Stato è chiamato a dare del suo e questo disegno di legge, voluto dalla Lega e a prima firma dell'onorevole Caparvi, prevede di muoversi lungo due direttrici, razionalizzando e mettendo a sistema i tanti eventi rievocativi di vicende e momenti del passato presenti sul nostro territorio, ma prima ancora selezionando e certificando gli eventi di qualità sicura dai tanti che non rispondono ai requisiti minimi di credibilità e scientificità. La qualità si misura, in questo caso, dalla fedeltà alla storia, dall'uso di linguaggio e costumi pertinenti all'epoca storica, in una parola dalla coerenza di quanto rappresentato con ciò che è realmente accaduto. Occorre, in altre parole, che gli eventi siano rievocati al di fuori delle mitologie e delle false interpretazioni, pur accumulatesi nel tempo. Questa qualità intrinseca di un evento di questo tipo, misurata sull'attendibilità e fedeltà scientifica delle rievocazioni, oggi è, fra l'altro, minacciata non solo dalla superficialità e dalla incultura dominante, ma anche da quella pervasiva ideologia che si ripromette non solo di cancellare, ma anche di riscrivere il passato, secondo canoni attuali o astratti spesso politicamente orientati. È chiaro che solo i primi andranno promossi e valorizzati, secondo l'insindacabile giudizio di un autorevole comitato tecnico scientifico, che la legge oggi alla nostra approvazione prevede e che, anzi, costituirà il motore che la metterà in moto. Ugualmente, proprio per meglio razionalizzare l'opera di promozione degli eventi di rievocazione storica più significativi, la legge prevede l'istituzione di un albo degli eventi e degli enti promotori riconosciuti. Al comitato, quindi, spetterà ogni anno di rendere nota la tabella degli eventi accreditati, mettendo a disposizione di enti, fondazioni, industrie e privati, uno strumento indispensabile per un'operazione di promozione sinergica degli stessi. La ricaduta in termini turistici, industriali e di coesione sociale e di riconoscimento, da parte di ogni territorio, della propria identità storico-culturale specifica sarà così facilitata. Il disegno delega, altresì, il Governo ad adottare norme per la salvaguardia del patrimonio immateriale nell'ottica delle direttive UNESCO e dei trattati firmati dal nostro Paese. Quindi, a nome del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, da sempre impegnato nella promozione e valorizzazione delle tradizioni locali e dell'identità dei nostri territori, dichiaro quindi, con convinzione, il nostro voto favorevole al disegno di legge.

ma origina da due proposte diverse: una disciplina la materia, appunto, delle rievocazioni storiche, su cui forse davvero sarebbe bastata un'iniziativa ministeriale; l'altra è una delega al Governo per l'emanazione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che non può, appunto, limitarsi alle manifestazioni di rievocazione storica. Forse, aver messo insieme questi testi rischia di essere fuorviante o limitante per il concetto di patrimonio culturale immateriale, perché, a parte un più visibile patrimonio costituito da eventi, scadenze, feste e riti, il patrimonio culturale immateriale allude a saperi, tecniche, espressività, legate anche a dimensioni familiari, sociali e lavorative dei diversi contesti. emerge attraverso la ricerca e la costruzione di rapporti di collaborazione e di alleanza tra ricercatori e attori sociali. Gli attori sociali sono molto importanti nella costruzione della dimensione del patrimonio immateriale come qualcosa di vivo.

articolo 8, che noi non condividiamo, il quale regola il porto e l'uso di armi in occasione delle manifestazioni. Pensiamo non sia necessario questo intervento di modifica della legge sulla detenzione e la raccolta delle armi da guerra, per cui è previsto il divieto. Sul patrimonio culturale immateriale, invece, pensiamo sia necessaria una normativa organica. È un senso anche di un salto culturale che noi dobbiamo fare, come Paese, di un'attenzione alla diversità culturale, anche di fronte, anzi, soprattutto di fronte ai fenomeni di globalizzazione. Questa attenzione alla diversità culturale aiuta il dialogo interculturale e il rispetto reciproco dei diversi modi di vivere. Fa scoprire somiglianze, tratti comuni, anche tra culture molto diverse. Quindi, è tutto il contrario della chiusura dentro il locale. La sua importanza risiede non nella manifestazione culturale in sé, ma nella ricchezza di conoscenze e competenze che vengono trasmesse da una generazione a un'altra. Questo è il senso anche della Convenzione dell'UNESCO del 2003, che abbiamo ratificato nel 2007. Tuttavia, proprio perché

culturale, che associa bene culturale a eredità: il bene non è assoggettabile al concetto di proprietà. L'elemento candidabile a essere bene immateriale rappresenta, appunto, la diversità e la creatività umana. Deve possedere possedere caratteristiche vitali; per l'Italia, ad esempio, parliamo dell'opera dei pupi siciliani, del canto a tenore sardo, della dieta mediterranea. codice dei beni culturali si è adeguato, ma fino a un certo punto, perché il salto di qualità consiste nel far uscire davvero le tradizioni dai libri e dai musei, in cui sembravano confinate, e nel far emergere la storia di memorie orali, oggetti folclorici, tracce vive di storie subalterne e spesso marginalizzate, che chiedono riconoscimento. Esse sono venute fuori anche grazie all'impegno di intellettuali e studiosi. È una vera e propria «comunità di eredità»,

i nuovi criteri per il fondo che finanzia i piccoli musei, che rischiano di penalizzare proprio le realtà più piccole, che spesso sono la soglia di accesso a questo patrimonio immateriale e raccolgono le tradizioni di una comunità. infatti innalzato il limite di bilancio di questi musei a 50.000 euro e il finanziamento fino a 100.000 euro, rischiando di perdere quel finanziamento diffuso che animava anche questi musei. Il patrimonio immateriale non è materiale, ma spesso in questi musei si trova il luogo di costruzione della comunità. Penso al Museo di comunità Remiero, che parla della cantieristica navale. Stiamo parlando di saperi molto vari, basati,

che i testi prendano atto, per una cultura che non guardi tanto alla specificità e all'eccellenza, quanto alla salvaguardia delle diversità e della vitalità delle comunità. Per questo noi pensiamo che i decreti attuativi di questo disegno di legge delega, che comunque voteremo, debbano essere condivisi e discussi con le comunità, con i soggetti, con le università, Operiamo uno spostamento dall'oggetto al soggetto della cultura, dagli oggetti alle pratiche e alle persone. Non si può fare patrimonio dei beni immateriali senza popolo, senza cittadinanza attiva, senza competenze ed esperti, che per questo motivo noi chiediamo vengano coinvolti. Dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico. Presidente, onorevoli colleghi, oggi ci troviamo a discutere una proposta di legge fondamentale per la salvaguardia della storia e delle tradizioni del nostro Paese. Le disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, contenute in questa proposta di legge di iniziativa del collega Mollicone, che arriva in quest'Aula dopo la prima lettura della Camera e dopo un attento esame in Commissione qui al Senato, sono disposizioni necessarie per mantenere vivo e tutelare il cuore pulsante di moltissimi territori, di moltissimi piccoli centri, ovvero di moltissime tradizioni. Si tratta di quel patrimonio materiale e immateriale di cui il nostro Paese è straricco. legge mira non solo a preservare, ma anche a valorizzare il Made in Italy, il marchio di eccellenza riconosciuto in tutto il mondo. Il Made in Italy rappresenta un simbolo di qualità, artigianalità e innovazione. Le nostre tradizioni, i nostri prodotti, il nostro patrimonio culturale sono il frutto di secoli di storia e di un sapere tramandato di generazione in generazione. Le manifestazioni di rievocazione storica, infatti, sono un esempio tangibile di come il passato possa vivere nel presente, offrendo un'esperienza unica e autentica sia ai cittadini che ai turisti. *(Applausi)*. Il Parlamento ha finalmente una particolare attenzione alla cultura e a questa problematica che ormai era imprescindibile sanare con il dettato contenuto in questa norma. Infatti, si ha l'obiettivo di definire le competenze dello Stato e della Conferenza unificata e di istituire un comitato tecnico-scientifico che dovrà chiarire anche un panorama italiano molto variegato, perché alle volte si può commettere l'errore di definire rievocazioni storiche anche quegli eventi che, benché abbiano il loro seguito e la loro importanza, non basano la propria natura direttamente su una ricerca storica puntuale. modo, si può fare l'errore di considerare rievocazioni storiche quegli eventi che si ripetono da secoli, ma che di fatto - poi - non sono rievocazioni storiche, bensì sono continuazioni storiche. un cambio di paradigma atteso da tempo, come la definizione di ciò che è patrimonio culturale, che va oltre la definizione dell'articolo 7-*bis* del codice Urbani, introducendo una inconsueta, ma necessaria iniziativa legislativa. l'UNESCO ha già accordato la necessità di affiancare l'importante patrimonio immateriale, che ha pari dignità ed estrema connessione, al patrimonio materiale e con il lavoro fatto con l'esame di questo provvedimento e la sua approvazione oggi possiamo finalmente definire che sono imprescindibili entrambi. Il codice Urbani andava definito in modo da avere una legge chiara che non lasciasse margini a interpretazioni, ma soprattutto che iniziasse a dare spazio e fattibilità, oltre che l'attesa dignità, a tutto quel patrimonio immateriale che a oggi non era considerato. Infatti, finalmente eguagliamo e soprattutto definiamo che il patrimonio culturale materiale non è tale senza la sua dimensione immateriale, senza sapere ciò che esso rappresenta, la sua funzione storica, culturale e sociale. Per questo, la legge che oggi votiamo contribuisce in maniera sistematica alla salvaguardia delle manifestazioni e degli enti di rievocazione storica. La trasmissione da una generazione all'altra di una tradizione porta con sé la possibilità che alcuni elementi del patrimonio culturale immateriale vadano estinti. La salvaguardia entra in campo quanto vi è qualcosa da tutelare. L'Italia è un patrimonio immateriale esteso e conosciuto. Questa legge e la sua definizione serviranno a tutelare - sì - quello già esistente, ma soprattutto a sostenere l'evoluzione del patrimonio culturale immateriale stesso, perché per noi è in continua crescita e continuo movimento. Le nostre comunità muovono e smuovono il patrimonio immateriale, sono loro a tutelarlo, sostenerlo e accrescerlo. È l'identità che entra e fa la storia. Basta citare la Convenzione dell'UNESCO del 2003: per patrimonio culturale immateriale si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni e le conoscenze, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questa definizione veste a pennello la nostra Italia, i nostri paesini e i nostri borghi, in cui vivere sembra essere un modo per dire di essere fuori dal tempo e dalla storia. Rievocare vuol dire, invece, ridonare tempo e storia anche a quell'Italia che non è un'Italia meno importante, produttiva o evoluta. Io sono nata in uno di questi territori, a San Nicandro Garganico, un piccolissimo Comune della Provincia di Foggia. Vi è tantissimo patrimonio immateriale da salvaguardare perché sono luoghi belli da vivere, belli da visitare e rappresentano l'identità nazionale e uno strumento di diffusione della conoscenza della storia italiana in Europa e nel mondo. La Regione Puglia, in particolare, è un esempio straordinario di come le tradizioni possono essere preservate e valorizzate. Le rievocazioni storiche pugliesi come la famosa Disfida di Barletta, non solo celebrano eventi storici significativi, ma promuovono anche il turismo culturale e l'economia locale. Io stessa ho presentato una proposta di legge sul valore degli abiti storici, sulla manifattura e sulla cura dei materiali. Ci sarà, una volta approvata alla Camera, una Giornata nazionale degli abiti storici, occasione in cui molti Comuni possono approfittare dei fondi messi a disposizione per organizzare convegni, manifestazioni e *workshop*. Gli abiti storici, realizzati con cura e attenzione ai dettagli, sono veri e propri capolavori della sartoria italiana che riflettono la ricchezza e la diversità del nostro patrimonio culturale. Inoltre, sono un elemento fondamentale delle rievocazioni. Ogni costume racconta una storia e rappresenta un'epoca e un contesto sociale specifico. Questi abiti non sono solo vestiti, ma veri pezzi di storia indossabili, che ci permettono di rivivere il passato e di comprendere meglio le nostre radici. La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è essenziale per mantenere viva la nostra identità. Le rievocazioni storiche non sono solo spettacoli, ma momenti di riflessione e di educazione che ci aiutano a comprendere chi siamo e da dove veniamo. Attraverso questo disegno di legge vogliamo garantire che queste tradizioni possano continuare a essere tramandate e che il nostro patrimonio culturale immateriale sia protetto e valorizzato. Votare questa proposta di legge contribuisce ad un passo importante per la tutela e la promozione delle nostre tradizioni, del Made in Italy e del patrimonio culturale immateriale. Insieme possiamo garantire che le future generazioni possano continuare a godere della ricchezza e della bellezza della nostra storia e della nostra cultura. Per questo e per tanto altro ancora, esprimo il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

siccome non possiamo lasciare nel Resoconto un riferimento a dati non corretti, perché non lo trovo corretto, mi vedo costretto, mio malgrado, a correggere la senatrice Aloisio, che ha fatto riferimento a una cifra irrisoria di 10.000 euro che sarebbe destinata alle rievocazioni storiche. Non è così, senatrice Aloisio, perché esiste la legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 627, che stabilisce

Presidente, è piuttosto inusuale che il Governo, alla fine degli interventi in dichiarazione di voto, intervenga per chiosare gli interventi delle dichiarazioni. A questo punto le chiedo, alla luce delle dichiarazioni del Governo, che si riapra la discussione. Senatore Borghi, le confermo che se il Governo interviene dopo le dichiarazioni di voto, si possono riaprire le dichiarazioni. Cito il comma 2 dell'articolo 99 del Regolamento: «Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento (…), prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, cinque Senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare». *(Commenti)*. Quindi, vi chiedo se ci sono interventi, altrimenti procediamo con il voto.

dei precedenti fondi già esistenti, che però venivano definiti assolutamente molto scarsi. Pirondini, ha facoltà di intervenire, se vuole, per un'ulteriore dichiarazione, come previsto dal Regolamento, altrimenti si procede con il voto. Volevo sottolineare che forse il Sottosegretario non ha sentito bene l'intervento che abbiamo fatto, perché è stato fatto un richiamo specifico a fondi che già già esistevano, che sono quelli che lei ha citato, ma che noi abbiamo definito scarsi, ai quali si aggiungevano la cifra che la senatrice Aloisio ha specificato. Quindi, per la prossima volta, il consiglio è prima di intervenire prima del voto, di ascoltare meglio gli interventi che poi si vanno a contestare in modo errato, come lei ha chiaramente fatto oggi.

di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. La 7a Commissione

Presidente, colleghe e colleghi, stupisce e ci preoccupa l'opera di disinformazione a cui si sta assistendo in merito alla ricerca sui giovani *gender variant* dell'Università degli una speculazione a cui stanno contribuendo anche diversi esponenti della maggioranza. L'università in questione, rinomata per la sua solida reputazione scientifica, ha precisato in un comunicato stampa che lo studio è una ricerca scientifica di natura qualitativa, focalizzata sul benessere di bambini, bambine e adolescenti con espressione e/o identità di genere non normativamente riconosciuti dall'Organizzazione mondiale della sanità. L'obiettivo è approfondire il loro vissuto emotivo e le dinamiche di relazione in ambito familiare e scolastico, al fine di tutelare i loro diritti. Si è tuttavia scatenato un violento attacco contro il gruppo di ricerca dell'Università Roma Tre e, nonostante questo lavoro fosse stato approvato dal comitato etico dell'ateneo, è stato preso di mira da alcune associazioni che hanno diffuso informazioni errate, articoli fuorvianti e condotto campagne diffamatorie sui *social.* Queste associazioni hanno inoltre divulgato i nomi dei ricercatori, esponendoli a campagne d'odio e seminando paura tra le famiglie che avevano partecipato volontariamente alla ricerca. credo che tutto questo sia molto grave e che violi totalmente la libertà di ricerca, oltre al fatto che non è mai corretto attivare una vera e propria macchina del fango. Esprimo pertanto la mia piena solidarietà ai ricercatori, alla direttrice del dipartimento di scienze della formazione e al rettore dell'Università Roma Tre e, ovviamente, alle famiglie che si sono trovate sotto attacco; signora Presidente, che, insieme all'università, hanno come unico obiettivo il benessere dei loro figli e delle loro figlie. Su questo ci dovremmo concentrare tutte e tutti, anziché sprecare energie ad arginare polemiche strumentali e crociate ideologiche.

di intervenire su scelte libere di chi fa ricerca, perché la ricerca è libera e per sua stessa natura (signora Presidente, so che lei sa benissimo cosa significhi fare ricerca) va a indagare ciò che oggi non è indagato, per conoscere

piacciano o meno, ci sono e che per ora sono state indagate solo nella fascia dell'adolescenza e non dell'infanzia, sulle quali non si intende intervenire in chissà che modo, ma portando avanti l'ascolto che la pedagogia,

di quello che questa università ha fatto per mettere in evidenza davanti a tutti che questo Governo non ha nessuna intenzione di toccare la ricerca libera ed è a fianco dei ricercatori di tutto il Paese.

tramite *social* e *mail* che si sono riversate nei confronti del Rettore, che stava semplicemente garantendo lo svolgimento del compito principale di un'università, che è quello della ricerca affiancato alla didattica, come hanno ben espresso le mie colleghe. Tutto questo, nella scia di una furia oscurantista che sta imperversando nel nostro Paese e i versi animaleschi che si levano dai banchi della destra non fanno altro che dimostrare la correttezza delle mie affermazioni. il mondo *pro* vita e *pro* famiglia dovrebbe guardare con interesse a questo genere di ricerche perché, visto che non fanno altro che proclamare continuamente che le disforie di genere non esistono, che sono tutta un'invenzione dell'ideologia *woke*, dovrebbero guardare con favore a ricerche che potrebbero supportare questa loro tesi. Se invece si scagliano con tanta furia contro la ricerca libera e il diritto di ricerca all'interno delle nostre università, forse è perché sanno che la negazione delle disforie di genere, è - quella sì - un'ideologia oscurantista e medievale che è nelle loro teste e quindi si ribellano contro la ricerca perché potrebbe esclusivamente dimostrare che la disforia di genere esiste, che è un dato di fatto e che continuare a negarla non può che far male ai nostri bambini, ai nostri adolescenti e alla nostra società che guarda al futuro e non al passato.

si pretende di piegare l'oggettività della scienza a questioni ideologiche, questo è sempre molto preoccupante, perché la scienza dovrebbe essere una sorta di stella polare che va al di là delle posizioni ideologiche (la mela che cade sulla testa di Newton - la forza di gravità - quella è, non è di destra o di sinistra) e noi dobbiamo essere interessati perché perché vogliamo portare avanti il nostro Paese, vogliamo sapere che cosa succede nel mondo della realtà attraverso gli occhi non ideologici ma pragmatici della scienza, perché questo ci dà strumenti per decidere nel nostro ruolo di legislatori. quindi, affermare che "le cose sono così" è sempre molto pericoloso, anche perché indebolisce la democrazia, in quanto dà meno strumenti di conoscenza a chi poi deve fare le leggi. leggi. Questo è preoccupante perché è portato avanti da una parte politica che davanti all'evidenza scientifica oppone una posizione ideologica e questo non rassicura per

colpisce un numero piccolo di persone, non per questo incide meno nella qualità della vita di quelle persone e delle persone che sono loro intorno. Credo quindi che dovremmo essere sempre attenti a cogliere tutte le opportunità che abbiamo per rendere quelle vite, che magari sono complicate, un po' più semplici. Chi decide di transitare da un genere all'altro, a qualsiasi età lo faccia, deve attraversare un'esperienza molto dolorosa: deve sottoporsi a interventi chirurgici, deve sottoporsi al biasimo e spesso alla violenza della realtà che ha intorno a sé. Se decide di attraversare queste fasi - la chirurgia, il dolore, lo stigma, la difficoltà di trovare lavoro e di relazionarsi in una società che non ha posto per te te - se nonostante tutto questo, queste persone fanno quel percorso, è perché la motivazione dentro di loro è talmente insopprimibile da portarle e portarli anche a sopportare tutto quel dolore. E allora, quando si attacca un'istituzione scientifica seria e prestigiosa come l'Università di Roma Tre, io credo che si faccia male tanto alla democrazia quanto

abbiamo appreso con assoluto sconcerto che un'università italiana stesse organizzando un laboratorio definito *gender creative*, un laboratorio sui ragazzini trans, perché l'università non è il luogo dove debbono essere svolti questo genere di laboratori, coinvolgendo minori.

a livello formativo dei nostri ragazzi sia altra e diversa. È per questo che abbiamo chiesto con un'interrogazione del vicepresidente della Camera dei deputati Rampelli di fare luce, avviando un'indagine sulla questione. Siamo sconcertati ogni volta che vediamo che nelle scuole di ogni ordine e grado si tende a svolgere corsi, momenti di quello che io chiamo in modo sereno indottrinamento dei nostri bambini che devono essere liberi di crescere senza forme alcune di indottrinamento di questo genere sul *gender* per poi, da adulti, scegliere quelle che sono le proprie inclinazioni. Tengo a ribadire che, come Gruppo Fratelli d'Italia, speriamo venga fatta presto luce su quello che è accaduto in questa università

furia nei riguardi di queste forme di indottrinamento, che nulla hanno a che vedere con il benessere del minore che io credo invece tutta la comunità politica, trasversalmente, dovrebbe cercare di tutelare e salvaguardare.

e ricordare una persona che ha vissuto una vita esemplare, vista con gli occhi dei giorni nostri. Valter Brugiolo era quel bambino biondo che nel 1967 vinse lo Zecchino d'Oro cantando la canzone «Popoff» grazie a quella vittoria, venne guidato dalla sua lungimirante madre in un primo tempo a far parte del mondo della canzone, cantando con Gianni Morandi e

presiedette poi per anni questa scuola privata a lei intitolata. Però il passaggio storico che segna Valter Brugiolo è proprio legato alla canzone «Popoff». La canzone «Popoff» nel 1967 crea un momento di cesura rispetto ai tempi precedenti: ci fu un'Italia prima di Popoff e un'Italia dopo Popoff. Ricordiamo che era

una sorta di complesso di inferiorità che avevamo noi italiani nei loro confronti. In particolare noi bambini ci sentivamo un po' dei poveretti, mentre c'erano questi russi e questi americani, ma in questo caso i russi, "i cosacchi lunghi e fieri" che "a quaranta sotto zero se ne infischiano del gelo", mentre noi invece cercavamo il tepore delle nostre case. Ebbene, Popoff case. Ebbene, Popoff ci fece capire che anche i russi erano umani, perché, mentre i cosacchi resistono a quaranta sotto zero, lui rimane con lo stivale nella neve e resta fermo lì. Però a un certo punto anche i cosacchi si fermano per il freddo e lui invece, rotolando della neve, arriva al fiume Don, che ha anche un'importanza immaginifica fortissima per la nostra cultura comune, perché il fiume Don - ricordo - era il luogo dove ci fu il presidio alpino durante la Seconda guerra mondiale e dove avvenne la

Poi ci fu lo sfondamento di Nikolajevka e tornarono a casa. Ecco, con la canzone "Popoff" ci sentimmo tutti redenti e recuperammo questa nostra immagine e questa nostra autocoscienza rispetto al passato. Dopodiché ci fu il Sessantotto, ci furono i movimenti studenteschi e nacque l'Italia

Grazie